alla lettura da parte della senatrice segretario mi è parso di capire che la sintesi sia stata la seguente: a un certo punto della seduta, il presidente Matteoli chiede la sospensione;

Ora, siccome la questione è di indubbia delicatezza, chiederei di poter ampliare questa parte. Si è affrontato il tema di come discutere un bilancio dello Stato in assenza di un maxiemendamento pluriannunciato e mai depositato nella seduta di ieri che ci sia un minimo di particolari rispetto all'oggetto della discussione; credo che ciò abbia una sua importanza, altrimenti si svilirebbe il dibattito innescato dalle dichiarazioni del presidente Matteoli.

L'articolo 128 del nostro Regolamento, al comma 1, recita: «Gli emendamenti, di iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5ª Commissione permanente». Il comma 3 del medesimo articolo dice: «Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente». Ne consegue che gli emendamenti che non sono stati respinti in Commissione non possono essere presentati in Aula. 4 tuttavia afferma: «È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea», ed è questo il motivo per cui solitamente è consentita la presentazione di maxiemendamenti in Aula. Noi ci troviamo invece nella situazione in cui il testo pervenuto in quest'Aula dalla Camera, perché nessuna modificazione è stata introdotta in Commissione, visto che è mancato il voto di autorizzazione al relatore a riferire in Aula; e men che meno sono state apportate delle modifiche in quest'Aula, visto che non abbiamo ancora iniziato a votare. A questo punto, non essendo state introdotte modifiche né in Commissione né in Aula, che consentirebbero la presentazione del maxiemendamento in Aula, mi chiedo se sia ammissibile o no,

e il provvedimento venne approvato nella formulazione della Camera, senza la presentazione di emendamenti in Aula.

e che tanto più ci richiama, per il futuro, all'esigenza di creare le condizioni, anche di tipo regolamentare,

Anche però nella fattispecie che si sta determinando, cioè a Regolamento e a legislazione vigente, la mia opinione è che la questione posta dal vice presidente Calderoli debba essere affrontata nei seguenti termini. Effettivamente, un problema di ammissibilità si porrebbe per quelle parti, da individuare, del maxiemendamento presentato dal Governo che non richiamino esplicitamente o implicitamente, cioè con riformulazioni, le materie affrontate dagli emendamenti presentati in Commissione, tutti gli emendamenti presentati. Sostenere Sostenere la tesi opposta equivarrebbe ad affermare che, se la Commissione bilancio non conclude i suoi lavori, non è apponibile la questione di fiducia sul testo della legge finanziaria. È evidente che questa conclusione prova troppo o si

La mia opinione è che questa interpretazione sia legittima, ma indubbiamente non corretta. Credo invece

per verificare se il Governo non abbia introdotto nel testo del maxiemendamento norme completamente avulse dai testi all'esame della 5ª Commissione.

È chiaro che non si può andare ad un riscontro testuale, ma è essenziale che una questione

così, travolgeremmo la norma del Regolamento del Senato a cui faceva riferimento il vice presidente Calderoli che, invece credo dobbiamo rispettare. Quindi

lo leggeremo - che il Governo abbia introdotto norme completamente nuove e non affrontate in emendamenti presentati in Commissione bilancio. In quel caso, a mio giudizio, bisognerebbe andare a una dichiarazione di non ammissibilità; in tutti gli altri casi ritengo che si debba sostenere l'ammissibilità del maxiemendamento, trattandosi, in caso contrario, di sostenere qualcosa di evidentemente abnorme e cioè che, per definizione, se la 5a Commissione non finisce i suoi lavori, il Senato dovrebbe votare il testo dalla Camera così com'è. È evidente che ciò priva il Senato della sua capacità di intervenire e non credo che in tal senso lei, signor Presidente, potrebbe concludere. Naturalmente, non faccio il suo mestiere - per mia fortuna, nel senso che il suo è più oneroso e difficile del mio - però mi sono permesso, dal momento che prima debbo vedere il testo

Enrico Letta, a domanda dei giornalisti, rispose chiaramente che non era stato deciso di porre la questione di fiducia sul cosiddetto decreto Bersani, sul quale, invece, il Ministro venne a porla, al Senato, il martedì seguente. suddetta interrogazione è stata da me sollecitata ben cinque volte e la Presidenza del Senato mi ha cortesemente dato conto di averla a sua volta sollecitata presso il Governo. Quando

trova necessità nel voler difendere la prerogativa del Senato all'introduzione di modifiche rispetto al testo presentato. Noi riteniamo che ciò - come ha sostenuto il senatore Calderoli - venga espressamente

restringe il campo di applicazione delle prerogative per la presentazione degli emendamenti. La discussione che va svolta sulla finanziaria, pertanto, è *stricto iure*; e vi è un motivo, ossia obbedire alla legislazione che nel tempo si è succeduta e, quindi, alle leggi di contabilità,

frutto di una riflessione troppo veloce, schizofrenica e contraddittoria; il Parlamento, invece, deve avere i tempi e i modi di poterne esaminare, discutere e votare

che siamo stati messi in condizione di conoscere, ossia gli emendamenti presentati in Commissione, ma presentati al Senato. Qualsiasi altra formulazione (in aggiunta o in riformulazione) non può essere accettata come testo sul quale porre la questione di fiducia. Questo, non per volersi non per volersi attenere in modo eccessivo alle condizioni poste dal Regolamento, ma proprio perché verrebbero meno la necessità e la prerogativa del Senato di votare la fiducia su ciò che si conosce: non può dirsi conosciuto un argomento che non è stato trattato.

alle determinazioni che intende assumere. A me pare che ci sia un punto estremamente chiaro, riconosciuto dello stesso presidente Morando, cioè la fondatezza della questione posta dal vice presidente Calderoli. presidente Calderoli ha ricordato con grande chiarezza quello che prevede l'articolo 128 del nostro Regolamento, cioè quando si può verificare il caso di specie.

Infatti, ad esempio, oltre alla risposta che tutti siamo ansiosi di conoscere rispetto al pregresso decreto Bersani, sarebbe interessante sapere quando la fiducia è stata decisa dal Consiglio dei ministri e su quale testo, visto che non si è avuta notizia di convocazione del Consiglio dei ministri nella giornata odierna o di ieri sera. Si tratta di una questione sulla quale c'è un problema di correttezza di procedura,

pare rivendicare un potere di ammissibilità da parte della 5a Commissione, che è invece un potere della Presidenza del Senato. Su questo vorrei che si fosse estremamente chiari: è lei che si deve assumere questa responsabilità, Presidente, perché è lei che deve tutelare il diritto del Senato

ha scelto una strada che è quella di impedire il confronto parlamentare sul merito del provvedimento e di spostarlo sulla discussione politica sulla finanziaria, ricambiandola per la quarantacinquesima volta. Cosa diversa sarebbe stata se il Governo avesse depositato il maxiemendamento in Commissione bilancio, in modo tale che la Commissione bilancio avrebbe potuto verificarlo in termini di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ci sarà uno spazio in cui la 5a Commissione potrà deliberare sulla mancata copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione? Questa è una questione che pongo alla sua attenzione,

Ci dev'essere un passaggio in cui la Commissione bilancio abbia la possibilità di esprimersi sulla copertura finanziaria formalmente, non informalmente. È una questione di grande sostanza e ritengo che possa essere da lei data la risposta che credo sia dovuta.

la preoccupazione di un approfondimento su questo punto da parte degli Uffici del Senato l'ho avuta e quindi una riflessione è stata fatta. Noi abbiamo il dovere di trasmettere il maxiemendamento, su cui si pone la questione di fiducia, alla 5a Commissione per le questioni sulle quali è chiamata a darci il suo parere, ma sulla questione più generale non ho molti dubbi e vi voglio dire perché, cari colleghi. Non vi è dubbio - questa è la riflessione fatta all'interno della nostra struttura - che qualora il Governo si fosse limitato a presentare in questa fase un nuovo emendamento al disegno di legge finanziaria, la Presidenza avrebbe dovuto valutarne l'ammissibilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 128 del Regolamento. Ma è altrettanto chiaro che non è ipotizzabile un sindacato sul contenuto di un emendamento sull'approvazione del quale

ha carattere di assoluta priorità, perché da questa il Governo fa dipendere la propria sopravvivenza. Conseguentemente, la fiducia prevale sulle disposizioni regolamentari che disciplinano l'ordinario procedimento legislativo».

La Presidenza, peraltro, al fine di garantire all'Assemblea una migliore informazione in particolare sui profili finanziari dell'emendamento governativo sottoposto al suo voto, ne trasmette il testo alla Commissione bilancio

Se dovesse valere l'ipotesi che il Governo per porre una fiducia deve presentare qualcosa e sul voto di quel qualcosa può porre la fiducia, quel qualcosa dev'essere prima di tutto ammissibile e ne è testimonianza il fatto che il maxiemendamento viene trasmesso alla 5a Commissione. Quindi, non è che sia insindacabile, perché l'esame della 5a Commissione dovrà tenere conto delle coperture e della costituzionalità dell'emendamento presentato.

su un provvedimento e da alcuni precedenti, che non hanno a che fare, almeno per quanto mi risulta, con la vicenda in esame, abbiamo dedotto una conseguenza

dobbiamo sempre inserire questa vicenda nel processo legislativo, perché, se fosse vera la conseguenza che è stata adesso oggetto di quel

il provvedimento in esame; potrebbe prescindere dalle norme che presidiano, ad esempio, le procedure in materia di decreti-legge; potrebbe prescindere dalle norme che presidiano le procedure in materia di legge finanziaria. Se il Governo potesse fare tutto, noi nella legge finanziaria potremmo mettere tutto. Vi sono delle leggi che disciplinano questo settore così delicato, ma con la questione di fiducia il Governo supererebbe le questioni regolamentari, le questioni sostanziali forse, anche le questioni di copertura e questosarebbe il paradosso dei paradossi! Allora, Presidente, ritengo e mi auguro che quanto è stato dichiarato in quest'Aula rappresenti una riflessione e non una decisione, perché, se applicassimo tale risultato all'attività di quest'Aula, avremmo creato un precedente esplosivo, un precedente esplosivo, non solo per la finanziaria, ma per qualsiasi tipo di provvedimento, che potrebbe sganciarsi da qualsiasi sistema normativo

lui dimostrato in quest'Aula anche in occasione della presentazione della legge finanziaria, ancorché non come relatore, ma come Presidente di Commissione,

ma anche la maggioranza, il Governo e, soprattutto, l'opinione pubblica, che non deve leggere sui giornali norme delle quali non ha mai sentito parlare

Nella seduta del 2 febbraio 2006 questo problema fu affrontato dal presidente Pera con le seguenti parole: «Infatti» afferma il Presidente come rilevò la Giunta per il Regolamento nel parere del 19 marzo 1984 - la votazione della questione di fiducia ha carattere di assoluta priorità, perché da questa il Governo fa dipendere la propria sopravvivenza. Conseguentemente, la fiducia prevale sulle disposizioni regolamentari che disciplinano l'ordinario procedimento legislativo». Sono le parole di un Presidente del Senato, nemmeno legate ad un intervento di molti anni fa. *(Commenti dai Gruppi

dell'opposizione. Ho detto prima che, secondo me, avete posto un problema reale e pensavo che lo voleste voleste approfondire e discutere nel merito, senza una pregiudiziale polemica di parte, che io comunque sto cercando di non fare. Quello che adesso ha detto il presidente Marini ha al riguardo una decisione sul punto presa dal presidente Pera, che mi fa piacere sia presente, da me sollecitata.

apposizione della questione di fiducia su un testo di legge - non è importante quale - il problema, ineccepibile sotto il profilo regolamentare e costituzionale, che riguardava il fatto che, attraverso la procedura di voto che noi adottiamo quando su un testo di legge si appone la questione di fiducia, si poteva, anzi era ipotesi normale, ipotizzare che anche l'articolo 81 della Costituzione venisse completamente travolto. Come voi sapete, che quando viene apposta la questione di fiducia su un testo di legge da parte del Governo, essa prevale su tutto, prevale su tutto, tant'è vero che il nostro Regolamento non dà luogo all'esame preventivo sul disegno di legge, su cui si è messa la questione di fiducia, da parte della 5a Commissione, secondo la nostra prassi ordinaria.

depositato dall'Esecutivo, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia - «di consentirci una convocazione e una discussione che non si conclude con un voto, per la ragione che ho già spiegato». Il presidente Pera, esaminata la questione, prese una decisione di cui pubblicamente lo ringraziai allora e lo ringrazio anche adesso, ritenendo che fosse quella giusta, a Regolamento dato (anche se, secondo me, bisognerebbe cambiare il Regolamento, ma questa è un'altra cosa, adesso è ancora in gli dissi: «Lei dà un contributo importante per eventualmente far emergere problemi di scopertura di quei testi attraverso una discussione di cui il Presidente della Commissione bilancio darà conto». Signor Presidente, in una occasione molto importante, che alcuni colleghi ricorderanno, questa importantissima - sarà certamente una sciocchezza, però secondo me fu importantissima - decisione del presidente Pera diede luogo, come i colleghi ricorderanno (e lo ricorda certamente il Presidente, perché gli si propose un problema particolarmente delicato), ad una discussione nella Commissione bilancio che fece emergere decine di

e, adottando una soluzione che spero i colleghi ricorderanno, disse: «Signor Presidente, sul testo dirò quali parti

in maniera piuttosto piana - tieni conto dei problemi segnalati e cambialo nel senso di non determinare l'approvazione di una legge diffusamente scoperta dal punto di vista finanziario.

prendendo la decisione di sottrazione dal testo delle norme incriminate, soltanto quando il parere della Commissione era stato unanime, anche se non espresso con un voto, ma semplicemente con una discussione. Signor Presidente, non voglio far perdere tempo al Senato, ma non c'è dubbio che questo precedente ci dice che la decisione di conferire il testo è una decisione importante che dovremmo far seguire da una modifica regolamentare che renda la Commissione in grado di fornirle un parere. Vorrei dire al senatore Storace che non ho nessuna intenzione di sostituire il Presidente del Senato; mi sono limitato a dire se il Presidente vorrà adottare la prassi costantemente adottata dal presidente Pera, certo non mi sottrarrò all'impegno di convocare la Commissione e consentirò questa discussione, di cui darò conto puntualmente,

nessuna intenzione da parte mia di sostituirmi in un compito che, tra l'altro, è molto gravoso e che non ho alcuna intenzione di assumermi. Mi ero proposto, signor Presidente, di svolgere una funzione servente per lei, sostenendo che il problema posto dal vice presidente Calderoli esiste, ma non nel senso in cui lo interpreta il senatore Ferrara, il senatore Ferrara, il quale afferma che solo gli emendamenti di cui la 5a Commissione ha discusso possono essere oggetto dell'iniziativa legislativa contenuta nel testo dell'emendamento del Governo. Questo è chiaramente ultroneo. Io non ho detto questo. Ho detto che, secondo me, nel testo depositato dal Governo non ci debbono essere materie che non abbiano almeno un emendamento depositato in Commissione (non mi interessa se discusso o non discusso) da cui traggano la loro fonte di legittimazione ad essere presentate, appunto, come materie oggetto dell'emendamento del Governo. Senatore Ferrara, lei è un membro autorevole della nostra Commissione

in Aula sono inammissibili emendamenti che non siano stati presentati anche in Commissione. Ma se questo è vero, allora ha un senso proporci di esaminare

Presidente, vorrei rimanere sui problemi reali richiamati dal presidente Morando che mi trovano perfettamente d'accordo. Credo che per per decidere sia necessario conoscere, e allora noi dovremmo verificare il maxiemendamento annunciato e la sua complessità. Sulla base di ciò, pretendere che gli Uffici siano messi in condizione di valutare, comma per comma, il maxiemendamento del Governo, il quale deve essere accompagnato da una relazione tecnica, comma per comma. È questa la garanzia che vogliamo rispetto alla decisione di assumere per valutare adeguatamente la verifica delle quantificazioni e, soprattutto, l'ammissibilità sia rispetto alla copertura, sia rispetto ai contenuti propri. Vorrei accogliere l'invito del presidente Morando per una discussione e un confronto sereni e responsabili rispetto ad una questione di grande rilevanza, non soltanto soltanto ai fini del procedimento, ma perché stiamo parlando della manovra finanziaria, ne stiamo parlando a ridosso della fine dell'anno e abbiamo tutti una comune responsabilità istituzionale. Proprio per questo, non vorrei che fosse dispersa la riflessione del presidente Morando nel tentativo di individuare, al di là della lettera del Regolamento, un percorso che consenta di rispettare la dialettica tra Senato e Governo rispetto alla presentazione di un maxiemendamento che, sostanzialmente, riscrive il disegno di un'unica sottolineatura che vorrei evidenziare, presidente Morando. Signor Presidente, non ho seguito bene e tra l'altro approccio questo intervento con grande umiltà, ma credo che il riferimento che lei ha fatto (ho sentito che la data si

ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5a Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea». In sostanza, il senatore

il punto di interpretazione sul quale bisogna misurarsi e superare la lettera rispetto al buonsenso istituzionale e ad una corretta dialettica tra istituzioni

della fiducia che riguarda il voto, in merito al quale il Governo ritiene, su un provvedimento fondamentale, di legare la sua sorte. Se ragioniamo secondo queste coordinate, può darsi che riusciremo a trovare un percorso che consenta anche all'opposizione di esercitare, attraverso il ruolo e il lavoro della Commissione bilancio, il suo diritto-dovere

ma all'Italia, a tutti i cittadini e - non vorrei eccedere - alla sopravvivenza stessa del Parlamento. Vorrei, quindi, che lei richiamasse l'attenzione sul fatto che la Commissione bilancio

*(Ulivo)*. Il punto fondamentale adesso è quello di portare il Senato a conoscenza del maxiemendamento del Governo, dal momento che tale conoscenza avviene per altri canali, perché le agenzie di stampa dispongono di questo testo e ci sono abbondanti lanci uno di questi spero non sia fondato, perché la soluzione individuata per i *managers* pubblici, se fossero vere quelle notizie, sarebbe talmente risibile che pregherei il Governo di farne a meno.

credo sia propedeutico un atto importante e fondamentale, al di là delle considerazioni fatte ed in modo particolare riassunte dal Presidente della Commissione bilancio, il collega Morando, per le quali mi sembra vi sia ampia convergenza e condivisione. Il primo momento importante e qualificante, propedeutico al resto, è quello se lei, Presidente - perché questa facoltà è tutta della Presidenza - ritiene che gli argomenti argomenti contenuti nel maxiemendamento siano estranei o non estranei all'oggetto del documento, cioè alla finanziaria. Questo è un punto fondamentale e direi necessario. Quindi, sarà altresì necessario che lei abbia il tempo adeguato - non so se lo ha già avuto - per analizzare ed esaminare l'enorme numero e lo sappiamo sempre dalle agenzie di stampa - di commi che prevede il maxiemendamento per stabilire se vi sono materie che non hanno nulla a che fare e quindi si possono considerare estranee, così come in modo chiaro l'articolo 126-*bis,* al comma 2-*ter*, recita. Questo passaggio è fondamentale, altrimenti, la fiducia cadrebbe in una fattispecie di totale oscurità, dove il Governo potrebbe inserire tutto e il contrario di tutto e quindi, a prescindere dai contenuti, chiamerebbe a votare quel tutto e il contrario di tutto. Pertanto, signor Presidente, siamo convinti che ella vorrà svolgere appieno quanto di propria competenza e permettere poi il seguito, così come si sta delineando, riferendomi ancora una volta al presidente Morando, del percorso successivo.

Essendomi occupato di questi argomenti nella scorsa legislatura anche direttamente, devo osservare due questioni e avanzarne una terza che mi pare la logica conseguenza delle prime due. Innanzitutto, è corretta la ricostruzione dei fatti e della genesi della procedura, relativa all'invio in Commissione bilancio dell'emendamento sul sul quale il Governo pone la fiducia, fatta dal senatore Morando: è andata esattamente nei termini da lui si era già evidenziato in quella sede come non soltanto la copertura, ma anche l'assoluta novità rispetto al lavoro di Commissione o agli emendamenti presentati in Commissione, fossero censurabili. La cosa si è andata evolvendo, perché in una di quelle leggi, esattamente sulla base di queste censure, in particolare con riferimento all'articolo 81, il consenso del Governo, per non violare il primato dell'Esecutivo nell'apposizione della questione di fiducia, espungemmo era stata posta, decine di commi, soprattutto perché erano scoperti, ma anche perché alcuni di essi affrontavano questioni totalmente sconosciute al lavoro fino a quel punto svolto.

La seconda questione riguarda un approfondimento che volevo proporre, signor Presidente. Poiché la questione assume un carattere penetrante, allora

occupava i banchi di quest'Aula nella scorsa legislatura ricorda benissimo come allora, a parti invertite, le stesse questioni venivano toccate e si cercava

preliminari che in qualche modo ritardano - Presidente, parlerò pochissimo - l'atto formale di presentazione da parte del Governo del maxiemendamento. Sono cose che comprendo benissimo, però - mi rivolgo a lei, Presidente, e al ministro Vannino Chiti - non comprendo e non accetto l'improvvisazione di un Governo che, prima di depositare formalmente il maxiemendamento, si preoccupa non di venire nelle istituzioni, di seguire un dibattito e di rispondere a delle

del quale servirsi; lo ricordo al Governo e il Governo non dia nulla di scontato. Noi vogliamo che il maxiemendamento corrisponda al lavoro che è stato fatto in Commissione bilancio, per non vanificare sette giorni d'impegno effettivo che i senatori della maggioranza e dell'opposizione, guidati dal presidente Morando, hanno concretamente messo in campo. *(Applausi dai però, il rispetto del ruolo dei parlamentari, delle Commissioni e di coloro che hanno partecipato ai lavori, lo chiede un senatore della Repubblica, dovrebbe pretenderlo dal Governo il rappresentante di tutti noi: la Presidenza del Senato.

noi non ci scandalizzeremo più di tanto se il nuovo testo sarà differente dagli emendamenti proposti: ciò fa parte delle competenze e delle possibilità del Governo.

Calderoli non ha posto un problema di esame e valutazione dell'atto, non si è fatto carico di questioni di merito. Signor Presidente, è stato evocato in quest'Aula l'articolo 128 del Regolamento ed ognuno, dal proprio punto di vista, ha detto cose

la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi». Quindi, non può essere nessun altro che lei. Si tratta di un problema al quale mi sono affezionato; credo che ritornerò, anche in modo informale, a discuterne con lei, però, la prego, signor Presidente, non si facciano evocazioni di casi precedenti in quest'Aula. Entro in quest'Assemblea in questa legislatura, per me esiste il diritto positivo, il diritto costituzionale e quello del Regolamento; non mi interessa il diritto materiale, io non c'entro con il diritto materiale. Ritorniamo al rispetto delle regole tutte, signor Presidente. Le riconosco, come già ho fatto per iscritto, di essere altamente sensibile e responsabile della necessità di tutelare le norme e i Regolamenti, quelli scritti. Pertanto, confido sulla possibilità

non possono essere ricompresi o che non abbiano un riferimento rispetto ai testi presentati in Commissione. Convengo su ciò e credo che sia giusto che si esprima un orientamento della Commissione, e lei, Presidente, poi deciderà come procedere.

a seguito dell'espressione della Commissione bilancio vengono stralciate le parti che non si attengono ai criteri prima stabiliti, e sul nuovo testo,

possiamo ledere il diritto costituzionale del Governo a chiedere la fiducia su un testo che esso ritiene legittimamente di presentare al Parlamento. Tale questione, Presidente, non può essere

a meno di 200 unità, non 200.000; immaginate se ciò fosse vero, ma lasciamo perdere. A me pare di registrare anche qui una scorrettezza, ma l'hanno fatto, molto meglio di me, colleghi anche della maggioranza:

per la storia della nostra attività, anche per l'applicazione del Regolamento. Signor Presidente, ho seguito con attenzione tutti gli interventi e mi ha colpito quello del collega Ripamonti,

in Aula di proposte emendative alla legge finanziaria non presentate in Commissione. Per me è sufficiente che le proposte fossero state presentate

che la Commissione bilancio sia deputata e investita in prima battuta e in maniera definitiva dell'argomento della finanziaria e di tutte le sue proposte di modifica. Il filtro necessario e indispensabile dell'Aula, pertanto, è la Commissione bilancio. Ma questo filtro, signor Presidente, allora vale per alcuni sì ed altri no? È questo il tema: noi riteniamo che valga per tutti, perché, ove così non dovesse essere, daremmo al Governo una capacità di penetrazione tale da irrompere nella rigidità dei Regolamenti parlamentari e da rompere un equilibrio che è fisiologico alla tutela infraparlamentare della nostra autonomia. *(Applausi dal

allora: vogliamo riconoscere al Governo questa ultracapacità di irrompere nei Regolamenti parlamentari attraverso il voto di fiducia e di presentare un emendamento nel quale, colleghi, si può parlare anche di altro, si può parlare anche di altro, di temi che non hanno nulla a che vedere con la finanziaria, con le leggi di bilancio e con l'ordinamento finanziario, perché si può parlare di tutto, di famiglia, di politica estera, se non vi è questo filtro?

un aumento del canone per le società di gestione degli aeroporti; trecento assunzioni di ispettori del lavoro; mille nuove agenzie. Signor Presidente, ci siamo ridotti a questo: ma la sovranità del Parlamento, dov'è?

adesso ‑ purtroppo e tristemente ‑ come Parlamento, dobbiamo abituarci a conoscere i contenuti delle proposte del Governo dalle agenzie prima che arrivino in quest'Aula: questo è molto preoccupante, è molto grave.

Il ministro Padoa-Schioppa non è mai venuto in Commissione bilancio; non so quante volte sia venuto in Aula (forse per il voto di fiducia); non abbiamo mai avuto il piacere e l'onore di averlo e di ascoltarlo, Venga il Ministro dell'economia a spiegare il senso di questa nuova manovra. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Abbia un sussulto di dignità e di coraggio per venire a spiegare qual è la proposta di questa sua nuova finanziaria: la illustri a quest'Aula!

quale è la nuova finanziaria. Non la facciano di nascosto, presentando un tomo di emendamenti, per poi approvarla con un violento, tempestivo e temerario voto di fiducia, durante la quale non si potrà che discutere all'interno di quest'Aula e non emendare alcunché.

ho molto apprezzato nella giornata di ieri il riferimento che il senatore Morando ha fatto al modo in cui si fa in Gran Bretagna la legge finanziaria: la mitica valigetta che viene portata in Parlamento, sulla quale si vota e non è possibile proporre emendamenti. Morando ricordava però che questo è preceduto da un intenso lavoro in Commissione, che dura due mesi e all'interno del quale la finanziaria è vagliata riga per riga. Quale è il sistema italiano? Teoricamente la finanziaria deve essere valutata dal Parlamento prima in Commissione e poi di nuovo in Aula; ammettiamo che è un po' troppo, ma questo è il sistema italiano: un sistema parlamentare con un doppio esame in Commissione e in Aula. Si conduce l'esame in Commissione, si impegnano nella Commissione, signor Presidente, grande energia, intelligenza, acribia; ci sono esperti di tutte le forze politiche di grande livello che si spendono nel tentativo di migliorare i provvedimenti. C'è dialogo tra maggioranza e opposizione per trovare, all'interno dell'impostazione politica della maggioranza, la possibilità di correggere errori e di migliorare qualitativamente i testi, fermi rimanendo gli orientamenti politici della maggioranza. Penso con amarezza, signor Presidente, al tempo che ho impegnato in questo lavoro, agli emendamenti che ho scritto. Penso con amarezza per me stesso, ma con assai maggiore amarezza per i colleghi della maggioranza che hanno impegnato intelligenza, amarezza per i colleghi della maggioranza che hanno impegnato intelligenza, competenza e capacità diplomatica e politica a trovare soluzioni che oggi affondano letteralmente nel nulla. E noi non abbiamo né l'esame in Commissione di due mesi, di due mesi, come in Gran Bretagna, né l'esame in Aula punto per punto, articolo per articolo; ci troviamo davanti non ad un emendamento, ma ad una nuova finanziaria. Una finanziaria che non verrà valutata da nessuno; una finanziaria davanti alla quale abbiamo un cambiamento della natura costituzionale dello Stato: altro che riforme istituzionali, altro che passaggio al sistema presidenziale. In nessun sistema presidenziale si propone una legge di bilancio o una finanziaria che il Parlamento deve votare o rifiutare praticamente senza conoscerla, perché per averne una conoscenza almeno sommaria, lei, signor Presidente, per difendere l'onore del Senato, dovrebbe sospendere i lavori, prendere una settimana di tempo e mandare in Commissione per una settimana il testo di questo maxiemendamento per poter fare finta di avere avuto un esame parlamentare e non per poterlo avere. Per poter credibilmente reggere la finzione che questa è ancora una Repubblica parlamentare, in cui vige la centralità del Parlamento e in cui non si è arrivati invece a qualcosa di assolutamente inedito: un Governo con poteri dittatoriali - qui sì veramente c'è una deriva plebiscitaria - che decide quello che crede,

Signor Presidente, la prego di prendere qualche iniziativa per difendere la natura democratica delle nostre istituzioni e la dignità di questo Senato. Presidente, questa discussione, come ha detto il presidente Matteoli, è stata sicuramente molto positiva per le due questioni che ha sollevato. Intanto la prima, di merito, sulla quale si sono cimentati gli esperti della materia. Abbiamo, di merito, sulla quale si sono cimentati gli esperti della materia. Abbiamo, infatti, ascoltato gli autorevolissimi Capigruppo della Commissione bilancio e tutti gli amici che si occupano di questa materia.

da una parte, messo un punto fermo, che nell'applauso generale dell'Aula ha significato una condivisione, e, dall'altro, aperto una riflessione che evidentemente non interessa solo la maggioranza o l'opposizione, ma tutti quanti di

che nel mese di gennaio, con il più largo concorso dei colleghi della Commissione bilancio stessa, avrebbe avviato un'ipotesi legislativa e di modifica del Regolamento del Senato per addivenire a qualche passo avanti nelle procedure e - perché no? - nei contenuti propri della legge finanziaria. Mi permetto di dire che sono totalmente d'accordo, che l'intero Gruppo dell'Ulivo è totalmente d'accordo, con la sintesi che può essere fatta sulla questione dal dibattito che si è svolto e che considero un patrimonio che viene offerto alla Presidenza

Poi, Presidente, si è aperta una seconda questione, sulla quale abbiamo ascoltato, con lo stile proprio dei protagonisti, diversi accenti. Parlo dei contenuti del maxiemendamento, delle procedure adottate, del rapporto tra Parlamento e Governo.

che il Governo, bianco, rosso o verde che fosse, ha posto la questione di fiducia, questi dibattiti sono stati più o meno sempre uguali. Essendo stato più volte protagonista di interventi più burrascosi e più polemici di quelli che sono stati fatti oggi qui, devo fare un apprezzamento ai colleghi dell'opposizione per il garbo, la profondità, la grinta e la serietà con le quali sono state poste le questioni

però, tutto questo bagaglio alle nostre spalle, dobbiamo anche eliminare gli eccessi di giudizi negativi su quanto sta accadendo.

Ora il Governo, alle ore 15 era qui per presentarlo, sono quasi le 17 e non glielo lasciamo presentare. Allora, siamo anche un po' contraddittori. Abbiamo detto più volte in questi giorni bisognava salvaguardare l'autonomia e la dignità del Senato, introducendo nel testo che veniva dalla Camera e sul quale il Governo aveva posto la fiducia, una serie di necessarie modificazioni. La Commissione bilancio ha operato e bene, con il concorso di tutti, per sette giorni e ha introdotto una serie di modificazioni in sede di Commissione. Infatti, colleghi, dobbiamo anche dire che fino all'articolo17 la Commissione bilancio ha approvato tutti gli emendamenti che riteneva di approvare, quindi non è vero che non c'è proprio niente, mentre sull'articolo 18 abbiamo dedicato un giorno all'illustrazione degli emendamenti e abbiamo anche un po' dialogato tra noi, quindi non siamo proprio a zero. E comunque, Presidente, il presidente Morando e tutti i Presidenti di Gruppo della maggioranza, devo dire insieme a quelli dell'opposizione, hanno più volte ribadito una loro aspettativa:

Abbiamo lavorato in Commissione e crediamo che sia giusto che il numero dei commi sia aumentato, perché chiediamo di integrare il testo venuto dalla Camera. In ultimo, Presidente, mi consenta di sottolineare che sulle procedure non ho parlato perché trovo l'interpretazione fatta da lei questo pomeriggio la più rispondente ad un'equa risoluzione della difficile e complessa interpretazione dell'articolo 128.

il maxiemendamento non è stato ricevuto. Noi siamo privi dell'elemento del contendere e lei, signor Presidente, se ce l'ha, ce lo dica, se non c'è l'ha, faccia come la Turandot, deve dire: «Il mio mistero è chiuso in me»! Lei lo deve dire, se ce l'ha o non ce l'ha Poi vorrei dire al ministro Chiti, che una volta ho scherzato e ho chiamato «il ministro Cheti», perché parla poco e quando parla è più «profondi silenzi ed altissima quiete»: fino a ora non ha dettoche cosa

avanti. È qui presente, dalle ore 15, il Ministro per i rapporti con il Parlamento con il testo del maxiemendamento.

per le determinazioni che dobbiamo adottare e che deve svolgere innanzitutto il Presidente con grande attenzione e senso di responsabilità, interpretando anche lo spirito di questo dibattito. Voglio

Alla fine, il rispetto delle prerogative e del ruolo del Parlamento passa da tante cose, ma anche da noi stessi, pertanto dobbiamo esercitare le nostre facoltà con grande attenzione. Comunico già da ora che appena il rappresentante del Governo

volevo porre questo problema. Alla luce, tra l'altro, della sua assunzione di un impegno su quella che dovrà essere l'attività della Commissione e sull'attenzione che lei assicura in relazione all'esito delle osservazioni che la Commissione elaborerà e - io dico - in relazione anche alla delicatezza del lavoro che la Commissione dovrà sostenere, volevo segnalare l'esigenza di dare alla Commissione ampio spazio temporale per poter realizzare questa attività. Non è infatti un'attività che si può svolgere nel giro di due o tre ore perché ci troviamo dinanzi un disegno di legge finanziaria in gran parte riscritto, non sappiamo con quali coperture sulle parti nuove e con quante parti nuove da espungere in quanto non oggetto di emendamenti presentati in Commissione. Ho voluto parlare prima che lei, signor Presidente, concludesse per, come si suol dire, mettere le mani avanti e dire: attenzione, noi dobbiamo consentire alla Commissione bilancio di poter lavorare in pienezza di autonomia, ma senza una costipazione dei tempi. Il nostro non vuol essere ostruzionismo (lei lo sa bene, signor Presidente; siamo stati sempre collaborativi in quest'Aula e addirittura a volte abbiamo chiesto la sospensione dei lavori per evitare di fare melina inutile nella consapevolezza di sapere che arrivava il maxiemendamento), non vogliamo assumere atteggiamenti ostruzionistici, però chiediamo che venga consentito alla Commissione bilancio di poter bene ed esaustivamente assolvere alle proprie funzioni su un tema così delicato e su una vicenda che si sta delineando così articolata e così complessa. Mi volevo permettere di ricordarle, signor Presidente, di non dare il programma all'Aula senza prima avere convocato

ma ha cercato di non ricordare ciò che molti senatori le avevano chiesto durante il dibattito: quando si esprime la Presidenza sulla estraneità di materia? Questo è un passaggio importante, altrimenti è inutile farci i complimenti a vicenda sul dibattito che c'è stato. Lei è stato richiamato - per carità, non ne aveva bisogno perché il senso di responsabilità che lei ha è riconosciuto da tutti e ancor più da me - prima dal me - prima dal senatore Calderoli e a seguire dal senatore Storace. Poi c'è stato un dibattito in quest'Aula partendo da questo presupposto. La Presidenza dovrà pronunciarsi e chiedo a lei quando intende farlo.

intervengo brevemente per allacciarmi alle osservazioni fatte dal presidente Schifani. A nome della Lega Nord Padania, volevo porre l'attenzione ulteriormente sulla questione dei tempi delle dimensioni prospettate del maxiemendamento e del lavoro della Commissione bilancio che, a questo punto, deve essere approfondito per permettere signor Presidente, di fare le valutazioni sull'eventuale necessità di espungere qualche norma che non sia conforme

Alla luce di questo, credo di poter anticipare quella che sarà la nostra posizione nella Conferenza dei Capigruppo che si riunirà

diano arbitrio ad un Ministro - il Ministro per i rapporti con il Parlamento - di decidere a suo piacimento che su un voto si gioca la vita del Governo.

porre la fiducia oggi ed è stato illustrato, nelle linee portanti e nel merito, il testo dell'emendamento; sono poi seguite le traduzioni tecniche e la relazione tecnica di accompagnamento. Non voglio con queste considerazioni fare polemiche o, almeno, non farne troppe, perché non è il momento e, francamente, non è neanche nel mio carattere. Tuttavia, al senatore Buttiglione - e

che da molti anni a questa parte la legge finanziaria, finché non cambia, chiunque sia al Governo e quale che sia l'ampiezza della maggioranza che ha il Governo, è ingestibile, se non viene purtroppo - aggiungo io - accompagnata da uno strumento come quello della fiducia? Se ve ne siete accorti, ritengo che questo sia il problema che dobbiamo in realtà affrontare, facendo in modo di non andare all'esercizio provvisorio

non governabile. Credo sinceramente, come abbiamo fatto noi in passato, che la Commissione bilancio avrebbe potuto concludere i propri lavori. Dico sinceramente che un tale atteggiamento anche negli anni scorsi avrebbe potuto determinare questa maggiore complicazione. Penso al tempo stesso

avrebbe potuto essere ancora più alto. Però, per sincerità e per correttezza, credo che una finanziaria così complessa e con tanti articoli - vi è una responsabilità anche

le considerazioni fatte alla Camera dal presidente Bertinotti, qui dal presente Marini, che il presidente della Commissione bilancio, senatore Morando, ha posto al centro del suo intervento in Aula, circa la necessità e di un impegno per cambiare lo strumento «legge finanziaria» e la sessione di bilancio già all'inizio del 2007. Per quanto riguarda l'emendamento presentato, esso scaturisce dal testo della Camera,

sarà distribuito. Ad esempio, la rivisitazione della norma sull'imposta di successione relativa all'impresa; gli incentivi alla rottamazione;

per il Veneto); una norma, che è stata approvata quasi all'unanimità (e quindi anche dall'opposizione), che modifica l'articolo 1 rimodulando la riduzione delle aliquote fiscali sulla base dell'incremento

Infine, sul problema dei conti dormienti è stata assunta la decisione, cui il Governo terrà fede, di accelerare la procedura di accertamento di quelli esistenti nelle banche,

alcune delle misure introdotte come novità nell'emendamento che il Governo presenta all'attenzione del Senato.

Penso che non sia normale e che non possiamo vivere con tranquillità la circostanza che per sei-sette mesi l'anno il Governo e il Parlamento siano occupati dietro la legge finanziaria

Il presidente Morando ha svolto considerazioni relative ai Regolamenti da modificare, alla legge di contabilità,

Camera, Senato, Governo, maggioranza e opposizione lavorassero attorno a queste modifiche, per avviare, come sottolineava il senatore Morando (credo sia un punto importante), un

Regioni e autonomie locali, a modificare per un altro aspetto la sessione di bilancio e i rapporti che si pongono a livello di Stato centrale, Regioni e autonomie.

solo una breve considerazione, anche perché l'intervento del Governo riapre in qualche modo il dibattito. Vorrei limitarmi ad osservare che l'esigenza di l'esigenza di ridisciplinare la finanziaria e la sessione di bilancio non può giustificare in alcun modo l'aggiramento o la mortificazione dei poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento. Lei, Presidente, si è impegnato a garantire comunque la discussione, anche nel caso di presentazione del maxiemendamento: questo sbarco dei mille, che or ora ci è stato annunziato, pur in assenza di Garibaldi che continua a latitare (mi riferisco al Ministro dell'economia).

di aver operato in tal senso, anche se è vero che, purtroppo, il maxiemendamento è proposto soltanto per permettere una minidiscussione, per di più priva di efficacia pratica.

di autorevolezza del Senato e dei suoi minimi indispensabili poteri di indirizzo e di controllo. Presidente, la prego di registrare ancora una volta il senso di responsabilità che l'opposizione sta manifestando. nel suo intervento il ministro Chiti non si è limitato a parlare della finanziaria e ad illustrare il maxiemendamento, ma ha affrontato anche problemi non inerenti alla legge finanziaria.

Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità l'organizzazione dei tempi di discussione della questione di fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria. Il testo dell'emendamento, corredato di relazione tecnica, è stato immediatamente trasmesso alla 5a Commissione permanente per la valutazione della copertura finanziaria, nel rispetto delle prerogative del Governo. Il Presidente della Commissione bilancio riferirà all'Assemblea in apertura della seduta antimeridiana di domani, il cui orario è stato posticipato alle ore 10. Avrà pertanto inizio la discussione generale sulla fiducia, che proseguirà fino alle ore 14 di domani mattina e quindi nel pomeriggio di domani, dalle ore 15 alle ore 22; nella mattinata di venerdì dalle ore 9 alle ore 14 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, per complessive 18 ore ripartite tra i Gruppi. Le dichiarazioni di voto finali, con trasmissione diretta televisiva, avranno pertanto inizio in ogni caso alle ore 18 di venerdì. Per cautela aggiungo che potrebbe esserci

L'Assemblea passerà poi, nella stessa serata di venerdì, dopo l'esame da parte della 5a Commissione permanente, alla votazione della Nota di variazioni al bilancio e al voto finale del bilancio medesimo, con la presenza del numero legale. Ove l'esame della Nota di variazioni dovesse protrarsi fino a ora tarda, la votazione del documento e la votazione finale del bilancio avranno luogo sabato mattina. Il Senato tornerà a riunirsi la prossima settimana in un'unica seduta, martedì 19 dicembre, alle ore 16, per il seguito dell'esame della legge comunitaria e per l'esame della ratifica della Convenzione UNESCO sulle diversità culturali fino a conclusione dei lavori.